«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza» (1452). Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia in sede deliberante con il parere della Commissione bilancio. Le predette Commissioni sono fin d'ora autorizzate a riunirsi per l'esame del provvedimento. **Sulle scritte offensive

fuori dai negozi e dai luoghi di culto che facevano parte di una cultura dell'odio. Ora crediamo che anche una cultura del politicamente corretto e della dittatura del politicamente corretto in qualche modo stia seminando

a questi esempi, a queste scritte e a questi messaggi che, ahimè, hanno avuto la storia e gli effetti che abbiamo conosciuto. *(Applausi)*. Prima di passare all'ordine del giorno, comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato all'unanimità alcune modifiche al calendario della prossima settimana e il nuovo calendario fino al 19 aprile. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di mercoledì 11 e nella giornata di giovedì 12 aprile per l'esame di ratifiche di accordi internazionali,

Nella settimana successiva il calendario prevede l'esame di mozioni sulla medicina di genere e sul *papilloma virus*, il seguito delle mozioni sull'industria agro-alimentare, il decreto-legge sul ripiano dei disavanzi nel settore sanitario quest'ultimo a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 18, con ripartizione dei tempi tra i Gruppi - nonché il seguito del disegno di legge per il riordino degli Enti di ricerca e un disegno di legge recante rideterminazione del termine di delega per il recepimento di direttive comunitarie. Le due prossime sedute pomeridiane del giovedì sono, come di consueto, dedicate al sindacato ispettivo; quella di giovedì 19 con particolare riguardo a materie di competenza del Ministero della giustizia.

finestra") *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci ritroviamo oggi a riesaminare il problema della violenza negli stadi, fenomeno che negli ultimi tempi sembra essere sfuggito di mano ai responsabili del settore, provocando sempre più episodi di violenza e di disordine, facendo apparire i nostri tifosi al resto del mondo come violenti, incivili e pericolosi e ogniqualvolta si svolga nelle nostre città anche la più piccola manifestazione calcistica è inevitabile che ci siano incidenti. Al fine di riottenere una certa credibilità, non solo nazionale ma anche internazionale, il Governo ha provveduto ad emanare un decreto-legge che colmasse in qualche modo i vuoti normativi che si sono venuti a creare nell'ultimo periodo, a causa della mancata applicazione del decreto Pisanu approvato nella scorsa legislatura. Il decreto-legge, dopo essere stato approvato all'unanimità al Senato, è ritornato dall'esame della Camera con evidenti profili di incostituzionalità e di disparità di trattamento e modifiche non condivisibili. Da un esame nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, sono stati rilevati dai colleghi senatori, sia di maggioranza che di opposizione, nonché dagli stessi relatori, diversi problemi. Mi riferisco in particolar modo alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 7 del decreto, in riferimento all'articolo 583-*quater* del codice penale, ove si è voluto affermare che per l'applicazione delle pene previste dalla fattispecie penale occorre che la circostanza lesiva al pubblico ufficiale venga procurata in occasione di manifestazioni sportive. Questo, onorevoli colleghi, è a dir poco scandaloso. Tutti noi componenti delle Commissioni 1a e 2 a, durante l'esame del decreto in questione, siamo rimasti a dir poco allibiti per come i componenti delle Commissioni della Camera dei deputati abbiano potuto modificare e approvare una norma tale da prevedere una evidentissima disparità di trattamento e non solo: con tale norma, infatti, si trasmetterebbe a tutta la popolazione un messaggio ambiguo che potrebbe far considerare tollerabili atti di violenza contro le forze dell'ordine in manifestazioni al di fuori di quelle sportive. Si potrebbe pensare, infatti, che nelle varie manifestazioni si possano commettere atti violenti contro le forze dell'ordine, con una diversa tutela per questi servitori dello Stato che molto spesso, specialmente nelle grandi città, sono continuamente a contatto con fenomeni violenti e di ordine pubblico. Fortunatamente in Commissione all'unanimità è stato deciso di richiedere le dovute modifiche all'articolo in questione, dimostrando, e di questo bisogna essere grati a tutti i componenti di maggioranza e di opposizione, un atteggiamento responsabile a modificare la norma.

Desidero evidenziare ancora la modifica apportata all'articolo 10, comma 1, capoverso 5-*bis*, del decreto in cui si configura nuovamente come una mera facoltà per le società sportive la partecipazione ai costi derivanti dall'adeguamento degli impianti sportivi ai requisiti richiesti dalle disposizioni normative. Anche qui le Commissioni hanno ritenuto di superare l'incertezza nell'individuazione dei soggetti competenti a provvedere agli adeguamenti richiesti ed è stato riproposto l'obbligo nei confronti delle società sportive di provvedere a tali oneri, anche per evitare che ulteriori spese gravino sui Comuni. Le società sportive pongano fine - lo diciamo con fermezza - agli stipendi *record* dei loro calciatori per finanziare una causa molto più nobile e sicuramente apprezzata da tutti i veri sportivi, utilizzando al meglio tali risorse per rendere più sicuri gli stadi. Un'ultima norma che desidero porre all'attenzione dell'Aula è quella relativa all'articolo 11-*ter*, in cui si prevede il rilascio di biglietti gratuiti nominativi per i minori di quattordici anni, accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado. Tale norma suscita diverse perplessità,

Presidente, sarò molto breve perché tutte le considerazioni che dovevamo svolgere le abbiamo già fatte questa mattina.

una parte del decreto che ancora non abbiamo approvato; una logica che sicuramente starà facendo rivoltare nella tomba Aristotele, ma tant'è. Vorrei sottolineare però alla presidente Finocchiaro, se ha la bontà

Ben venga, quindi, il risultato che si sta profilando per l'approvazione di un testo condiviso, rimandando l'ulteriore applicazione al disegno di legge già in discussione in Commissione. Già nel mio precedente intervento ebbi a dichiarare come tali misure siano auspicate e attese da moltissima parte della società civile e dagli sportivi italiani. Pertanto, mi onoro di partecipare al dibattito odierno con la convinzione di interpretare il sentire dell'opinione pubblica di un Paese, stufa di questa violenza fanatica e spesso politicizzata che sta devastando l'immagine del calcio italiano e minando i valori stessi sui quali si fonda lo sport. Il presente decreto-legge del Governo è da noi interpretato, e non potrebbe essere altrimenti, come la prosecuzione di un lavoro già avviato dal passato Governo, lavoro che si è tramutato in provvedimenti legislativi varati dal Parlamento nel corso della passata legislatura per contrastare la violenza nello sport. A dire il vero, colleghi dell'opposizione, allora il cosiddetto pacchetto Pisanu non incontrò, da parte vostra, la nostra stessa posizione costruttiva. Noi invece vi sosterremo, esprimendo al contempo il più vivo compiacimento per il ravvedimento che vi ha portato a superare la remore e le riserve del passato. Tali richiami al passato non sono per spirito di polemica, ma per controbattere a qualche affermazione che si è sentita e letta sulla stampa circa la mancanza di efficacia delle norme varate dal precedente Governo. Il fatto che si imputi oggi, anche da alcuni rappresentanti della sinistra, alla precedente legislazione la responsabilità di aver fallito nel contrastare la violenza, perché le norme varate allora erano troppo repressive, appare anche ai più sprovveduti una contraddizione in termini ed una cosa non rispondente alla realtà. La realtà è che quelle norme - che di repressivo avevano assai poco - sono risultate poco efficaci per la forte opposizione della sinistra, che si è impegnata a smontare le misure più efficaci ed ammorbidire tutte le altre. Il risultato finale fu che le leggi di quegli anni furono annacquate e, durante i dibattiti parlamentari, rese ancor meno efficaci per l'atteggiamento denunciato delle opposizioni. Oggi, dovendo correre ai ripari, la stessa sinistra che solo qualche anno fa non esitava a fare le barricate ci propone un provvedimento con misure più restrittive, le stesse probabilmente avverso le quali qualche anno fa, solo perché proposte dal Governo Berlusconi, non avrebbe esitato ad esprimere parere contrario bollandole come repressive e lesive della libertà. Ciò premesso, confermo il sostegno al presente testo, per giungere all'obiettivo di restituire gli stadi agli italiani, ai giovani, alle famiglie, ai tifosi, agli stessi *ultras*, quelli che vanno allo stadio - e sono la stragrande maggioranza - per vivere una bella giornata di sport. Il fatto che su questo ci sia una larga condivisione non potrà che rendere più forti ed efficaci le misure che ci apprestiamo ad adottare. Occorre comprendere, una volta per tutte, come tra i tifosi si celino delinquenti comuni che vanno allo stadio ma non guardano neppure la partita, considerano le tribune o le gradinate di una curva come il loro territorio, dove sono loro a dettare le regole, a comandare, e lo Stato ed i suoi rappresentanti sono visti come il nemico da offendere, da colpire, da allontanare e combattere. Un luogo dove sfogare la rabbia, esercitare la violenza, praticare la ribellione allo stato puro. Ribellione, in primo luogo contro le forze dell'ordine, che a Catania ha visto l'uccisione dell'ispettore Raciti e che a Livorno ha visto inneggiare a questo assassinio. E' chiaro che per questi soggetti il pallone, la partita, il tifo, è diventato solo un pretesto per esercitare la loro violenza, il loro potere: contro tali soggetti non è più possibile esitare. Condivisibili appaiono anche le misure auspicate a carico delle società, verso le quali, però, non potrà essere caricato tutto l'onere della responsabilità; sarà necessario mantenere alta la guardia e vigilare come istituzioni affinché non si arrivi, tra qualche anno, all'ammorbidimento di queste misure. Al riguardo vale la pena ricordare come in Inghilterra il fenomeno della violenza negli stadi è stato combattuto con impegno sinergico e costante, tra società, istituzioni e mondo dello sport. Un esempio può farci meglio capire come in Inghilterra sia riuscito questo intervento: negli stadi inglesi, durante le partite a rischio, è presente un giudice in grado di comminare pene in tempo reale ed immediatamente eseguibili. In conclusione, riconfermando quanto già delineato nel mio precedente intervento in quest'Aula, laddove già ci eravamo espressi positivamente riguardo alle nuove misure proposte dal Governo, ribadisco il massimo sostegno alle forze dell'ordine quotidianamente impegnate anche su questo fronte, con l'auspicio che da oggi il loro lavoro sarà più agevole ed efficace. *(Applausi

Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo, Insieme con l'Unione-Verdi-Comunisti Italiani, sosterrà con convinzione la conversione del decreto. Lo faremo con la consapevolezza, cui ho già fatto riferimento, che quello di oggi è un tassello che si deve inserire in un intervento più generale, volto a restituire dignità e valore alla cultura sportiva nel nostro Paese. Quello che oggi approveremo, spero con un consenso largo, è un provvedimento equilibrato, capace di introdurre, insieme a strumenti efficaci a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura, primi interventi di prevenzione e di promozione della cultura sportiva. È la dimostrazione di come un dibattito laico e sereno tra le forze politiche, unite da un comune obiettivo, e un'interlocuzione attenta e sensibile del Governo possano garantire la qualità che i cittadini si attendono. Siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo di battere la violenza siano necessari interventi complessi. Non vorremmo che, passata l'emergenza, i legittimi interessi e le diverse culture divengano un limite al linguaggio comune che oggi parliamo. Penso alla mutualità nella redistribuzione delle risorse legate ai diritti televisivi, o alla già citata proprietà degli stadi in capo alle società sportive. Ci auguriamo che questi temi verranno affrontati condividendo, come esito, la promozione della cultura sportiva e dei suoi valori, non la promozione solo della ricchezza delle società sportive. Un atteggiamento fondato sulla centralità del mercato non ha funzionato. Uno sport solo televisivo, fondato sulla competizione fuori dalle regole, in cui sia accettata un'impunità di fatto sarebbe un danno per il Paese, non una risorsa. Noi invece abbiamo l'obbligo di riaffermare i valori dello sport, non solo per un indistinto principio etico, ma per la consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte: uno sport malato produce e rafforza gli elementi di disgregazione sociale e funge da catalizzatore di forme di devianza sempre più aggressive. Intervenire nella scuola, ovviamente, diventa essenziale. Cogliamo già i primi messaggi in questo decreto, ma su questo terreno serviranno ulteriori interventi, specifici e puntuali, per restituire una centralità alla cultura sportiva nel percorso scolastico. Dobbiamo superare quella involuzione cui abbiamo assistito negli anni per cui l'ora di educazione fisica è un lungo intervallo e recuperare il valore forte dell'educazione sportiva. Non si tratta, come in tanti altri casi, di aggiungere pezzi all'orario scolastico, ma di restituire dignità ad uno spazio che già c'è per poi, casomai, aumentarlo. Ancora, importanti potrebbero essere le palestre, il luogo dove vanno milioni di amatori. Lo abbiamo denunciato spesso: oggi il mercato clandestino delle sostanze dopanti passa soprattutto per centinaia di palestre sporche. Promuovere lo sport pulito sarebbe un messaggio chiaro contro la cultura della vittoria a tutti i costi. Pertanto, proprio quando il primo tassello di questo *puzzle* viene approvato, è necessario ribadire come sia doveroso completare il disegno: un prossimo passaggio sarà la delega sui diritti televisivi, ma ci auguriamo di affrontare rapidamente anche gli altri aspetti di questa complessa problematica. Così come ci auguriamo che il clima di intesa che ha attraversato entrambi i rami del Parlamento possa proseguire. Quello che oggi approveremo, continuo a sperare con un consenso largo, è quindi un provvedimento equilibrato, capace di introdurre, insieme a strumenti efficaci a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura, primi interventi di prevenzione e di promozione della cultura sportiva. Ora tutta la società, nelle sue diverse articolazioni, deve mettersi al lavoro. Il mondo sportivo calcistico sta facendo la sua parte: dopo la guida saggia ed equilibrata del commissario Pancalli, succeduto al commissario Guido Rossi, a cui vanno i nostri complimenti, ieri è stato eletto presidente della Federcalcio Giancarlo Abete, a cui rivolgiamo i nostri auguri, il quale ha detto con chiarezza che nello sport l'etica è una precondizione e che non ci può essere sport se non c'è etica. Sono parole bene auguranti, per chi ritiene che l'autonomia dello sport e la cultura sportiva siano valori da preservare e custodire. E probabilmente il calcio deve anche ricostruire una credibilità negli ultimi anni troppo spesso minata. A partire da oggi, forze di polizia e magistratura hanno strumenti più efficaci per isolare i violenti. A noi legislatori, però, resta l'onere di completare l'opera. Lo dobbiamo non solo alla memoria di chi ha dato la vita, come l'ispettore Raciti e il dirigente Licursi, ma anche alle nostre forze dell'ordine, che garantiscono ogni domenica la sicurezza di tutti noi. Così come lo dobbiamo a quei milioni di tifosi che non sono violenti, per i quali la partita è la bellezza del gesto tecnico e non l'occasione per una rissa tra violenti. Signor Presidente, la Lega non può votare a favore di questo provvedimento per le motivazioni che abbiamo già illustrato e che vale la pena ripetere.

cosiddetto decreto Bersani. Ebbene, oggi credo che abbiamo raggiunto un bel livello, perché non soltanto siamo costretti a votare un provvedimento che non condividiamo in alcuni aspetti fondamentali,

Ci asterremo perché condividiamo invece la *ratio* della quasi totalità di quanto scritto nel provvedimento. Condividiamo il fatto che occorra dare un segnale forte a quei tifosi che non vogliono rassegnarsi a seguire le regole del vivere civile. Riteniamo quindi che questo sia un provvedimento che in qualche modo ci fa perdere un'occasione: l'occasione di varare

Dovremo seguire il destino che spesso ha la Lega: quando dice alcune cose non viene creduta e poi, dopo due o tre anni, si dirà che avevamo ragione. Questo sarà uno dei tanti casi, lo aggiungiamo alla lista.

impegnativa e significativa, ed è la ragione per la quale credo che il Gruppo UDC abbia concorso in modo rilevante a che questa stessa decisione sia presa oggi. Il Gruppo UDC voterà a favore della conversione del decreto-legge per come ci è stato trasmesso dalla Camera,

di fatto, di responsabilità nazionale, non è una decisione che riguarda questo Governo o i rapporti tra maggioranza e opposizione. È una decisione che il Senato prende in riferimento al generale mondo dello sport italiano, che aveva visto i gravissimi fatti di Catania come un punto di arrivo di un'evoluzione grave dell'illegalità diffusa nel contesto delle manifestazioni sportive del calcio italiano. Il mondo sportivo italiano ha in fondo accettato questo decreto‑legge che il Governo ha adottato, in continuità culturale con il cosiddetto decreto Pisanu, prendendo atto che in qualche misura vi poteva essere un cambiamento di clima da parte del mondo dello sport,

Questo è il fatto nuovo, la vera novità. Tutto il resto è molto opinabile. In quella sospensione delle partite di calcio vi è stata una decisione di straordinarietà legata alla vicenda catanese, e noi oggi assumiamo una decisione che riguarda questa straordinarietà. Votiamo a favore di un decreto-legge da convertire che scade tra pochi giorni. So perfettamente che è una decisione che ha un valore politico emblematico, ma è questo valore che ci ha portato una settimana fa a dare una soluzione possibile a questa vicenda: approvare il decreto come è, sapendo che le modifiche, se unanimi, da apportare in Commissione al Senato, devono diventare oggetto di un intervento del Governo nella stessa materia. Il Governo ci ha indicato che oggi non può, per ragioni costituzionali, adottare un decreto-legge nella stessa materia mentre questo è convertito. Si procederà allora con la sede deliberante presso le due Commissioni riunite. È una soluzione ragionevole. Confermo, a nome dell'UDC, il senso di responsabilità nazionale nel convertire questo decreto e mi auguro che questa nostra decisione

a rompere quel muro di reciproca incomunicabilità che vi è stato troppo a lungo tra il mondo dello sport - del calcio in particolare - e il mondo politico italiano. Lamento questa incomunicabilità come fatto grave per la cultura civile del nostro Paese.

Manteniamo la decisione del voto favorevole perché, come ho detto più volte, sarebbe impensabile lasciare per qualche tempo all'incertezza del voto finale della Camera un testo che, come tale, è atteso come segno di civiltà da parte del Parlamento italiano. In questo senso, lavoreremo di

intervenire ad adempiere a questi doveri; ebbene, alla Camera questa imposizione, questo dovere viene trasformato in facoltà. Noi siamo convinti che chi ha facoltà di poter non fare spese sicuramente non le farà.

non rilassiamoci in questi amabili conversari; vediamo di tenere l'attenzione più alta, in termini di silenzio e di ascolto.

la collaborazione del Governo, ma anche la lealtà di tutte le forze politiche che certo hanno condiviso questa strada subordinata per raggiungere lo stesso obiettivo. obiettivo. Di fronte a questa soluzione, pur ribadendo che la soluzione migliore era quella che avevamo prospettato, per il rispetto che abbiamo per le Forze di polizia, con la volontà di definire una rete normativa più severa nei confronti del ribellismo negli stadi, per il bene del mondo dello sport - di cui dobbiamo essere custodi

Ciò nonostante, pare che le ragioni della demagogia e della politica ci impongano di approvarlo immediatamente e di non affaticare, sia pure in questi giorni prepasquali, i colleghi della Camera per una rapidissima navetta e per l'approvazione di un disegno di legge forse più conforme ai nostri ordinamenti. So bene che il commissario Pancalli ha affermato che se oggi il Senato non dovesse approvare questo disegno di legge

dove erano quando quel mondo si è immarcito in ragione dei pesanti interessi economici che lo connotano e principalmente quando è stato silente in ordine ai perversi legami che spesso hanno collegato le società al mondo degli *ultras*.

mi chiedo, signor Ministro e signori colleghi senatori, se davvero ritenete giusto che chi provoca lesioni gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico debba rispondere di una pena particolarmente pesante se è tifoso, e invece di una molto più lieve nel caso in cui sia - che so - un attivista politico o un entusiasta di chissà quale forma di idea. Eppure, questa è la disposizione che vareremo lo faremo in piena lesione della nostra Costituzione. È infatti chiara la violazione dell'articolo 3, non essendovi ragionevolezza per questa disparità di trattamento, specie ove si pensi che la forma aggravata del reato di resistenza, che prevede addirittura una pena fino quasi a dodici anni, non fa distinzione fra le manifestazioni sportive e altro genere di manifestazioni. chiederà se il Presidente della Repubblica, che pure ha vigilanza e controllo sulla legalità costituzionale dei provvedimenti legislativi, firmerà o meno questo provvedimento: non mi interessa, non mi appartiene.

esponenti molto meno autorevoli di loro si erano permessi di fare in sede di Commissioni riunite. A fronte di queste chiare affermazioni, che non sono rimaste in un ambito salottiero ma sono state proclamate nell'Aula del Senato, mi domando come farà il Presidente della Repubblica a non soffermare, quanto meno, la sua attenzione sull'incostituzionalità o meno del provvedimento. Speriamo che non lo faccia,

Non debbo ricordare a voi come, in occasione della finanziaria, sia passato qui al Senato il comma 1343 perché non si poteva fare la navetta in situazione prenatalizia e voi siete stati costretti a presentare un disegno di legge per la modifica di quel comma, i cui effetti positivi o negativi sono devoluti all'attenzione della magistratura che si interesserà delle singole

per il varo di un provvedimento la cui scadenza è fissata al 9 aprile; ma come ho ricordato prima, probabilmente non si possono disturbare i colleghi deputati impegnati nelle ratifiche di qualche accordo internazionale, affinché

Il Governo, il ministro Amato, con tutta la sua autorevolezza e, devo dire, in piena sincerità, perché non ha taciuto le anomalie del provvedimento, ha chiesto al Senato di vararlo,

Noi aderiamo a tale richiesta, signor Presidente; non a caso, oggi stesso abbiamo consegnato in Commissione un disegno di legge attraverso il quale cerchiamo cerchiamo di modificare le anomalie che tutti voi avete segnalato in riferimento al provvedimento che di qui a poco approveremo. Certo è però, signor Presidente e signori senatori,

e impantanarsi alla Camera e non trovare la sua luce e il suo varo, per ottenere quelle modifiche che qui tutti noi abbiamo ritenuto giuste e corrette, comprese quelle scarsamente gradite alle *lobby* delle società di calcio, avremo

il grave atto istituzionale di considerare il Senato subvalente rispetto alla Camera dei deputati, forse avanzando una riforma costituzionale che qualcuno desidera, ma sicuramente andando contro la nostra Costituzione. Signor Presidente e signori senatori, ove mai si dovessero verificare ulteriori errori e i provvedimenti dovessero arrivare al Senato senza il tempo necessario per un loro corretto approfondimento, per una loro modifica e per un eventuale rinvio alla Camera dei deputati, più chiamarci al senso di responsabilità, perché voi siete la maggioranza, voi siete il Governo. Il vostro Presidente afferma che siete la serietà al Governo. E allora, se siete seri, cercate di sbagliare di meno; cercate di convincere, attraverso la simpatia della *moral suasion*, i vostri deputati e senatori a non commettere errori. Credo sia l'ultima volta che potrete richiamarci al senso di responsabilità ed è l'ultima volta che vi daremo una mano

potranno essere oggetto di lesioni gravi e gravissime da persone che non sono tifose, senza avere la necessaria soddisfazione di tipo giudiziario. Guardi, Presidente, chi conosce anche minimamente le questioni di diritto sa che la sanzione, oltre a modulare la pena

all'entusiasmo devastante e violento di diversi attivisti politici. Forza Italia voterà comunque a favore.

da una parte, la stringente necessità di dare una risposta seria e concreta ad una opinione pubblica che chiede ormai, da molte settimane, strumenti, iniziative, atti legislativi al Parlamento e, dall'altra, la necessità, emersa in maniera sufficientemente chiara, di rimettere mano al testo, di apportare una serie di importanti limature rispettando i tempi dell'approvazione. Non era facile, non è stato certamente facile; ma la strada che è stata tracciata dalla riunione congiunta tra Governo e Commissioni

delle attese non soltanto del mondo dello sport*,* ma più complessivamente dell'opinione pubblica nazionale. Credo che, al di là dei limiti del testo, cui sono convinto e siamo convinti si porrà rapidamente mano attraverso la Commissione e - credo di tranquillizzare in questo senso anche il senatore Castelli - le intese intercorse con la Camera, l'approvazione della legge sulla violenza nel calcio segni comunque un passo importante sulla strada della normalizzazione del tifo e, direi, più complessivamente dell'intero «sistema calcio» in Italia. Una legge, dicevo, lungamente attesa in queste settimane, inseguita con coraggio e passione da tutto il Parlamento; una legge che ha saputo costruire finalmente, caro Presidente, anche all'interno di quest'Aula una forte unità tra maggioranza e opposizione, confermando come lo sport non abbia bisogno di bandiere né di confuse ideologie, bensì di atti concreti, capaci di incanalare le sue enormi potenzialità, ma anche di frenare le sue inquietudini profonde. Tutti sappiamo, all'interno di quest'Aula, come questo atto rappresenti solo ed esclusivamente un primo momento, che chiude il sipario su quella che è stata una «terapia d'urto», una terapia di primo intervento che avrà bisogno non solo di adeguate correzioni, ma anche di essere, in futuro, monitorato costantemente e costantemente seguito. Tutti sappiamo come nei nostri stadi, dopo il dramma di Catania, il pallone non potrà rotolare più come una volta e questo decreto-legge, nelle sue proiezioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza, fotografa certamente una preoccupazione vera, determinando anche svolte autentiche, tutt'altro che formali. Una risposta che noi riteniamo forte, chiara, vera, autentica ad una situazione non più accettabile né sostenibile né sostenibile e che probabilmente, anche grazie all'applicazione più stringente del decreto Pisanu, può costituire una ricetta utile e possibile per il calcio italiano. Un altro calcio è possibile, ma bisogna (lo dicevo prima) monitorare costantemente, valutare, controllare controllare gli sviluppi conseguenti alle nostre iniziative legislative. Il calcio italiano viene da inquietudini profonde: Calciopoli è stata probabilmente l'ennesima realtà che ha toccato in maniera grave il nostro sport più popolare e direi complessivamente che questi mesi hanno messo a nudo in maniera chiara anche i limiti organizzativi, le oscure connivenze, i falsi luoghi comuni che hanno caratterizzato per troppi anni il rapporto tra società e tifosi e la complessa elaborazione del pianeta calcio. calcio. Credo che in questi anni la mancata applicazione di leggi esistenti, ma al tempo stesso il mancato inasprimento delle pene, abbia finito per determinare e per sviluppare una spirale assurda

Senatore Saporito, la prego, lei non smette nemmeno quando il Presidente raccomanda. di questa spirale assurda del calcio italiano, nella quale troppo spesso la parola «inedia» ha fatto rima con «tragedia». Ebbene, credo che oggi noi dobbiamo anche ringraziare il commissario Luca Pancalli, che ha lasciato il suo difficile e delicato compito, ha saputo confezionare in queste delicatissime settimane: una piattaforma coraggiosa, nuova, una trama diversa rispetto al sistema calcio che ha determinato indiscutibilmente anche difficoltà, problemi, implicite accuse verso il sistema calcio e verso la sua incapacità di uscire dalla spirale dei suoi equivoci, ma ha determinato soprattutto il segno di un cambiamento alto e forte del quale gli deve essere dato atto per l'impegno, per la dedizione e per la passione con la quale è riuscito ad inseguire questo obiettivo. oggi credo che dobbiamo salutare positivamente l'espressione pressoché unanime da parte della realtà calcistica nazionale del nuovo presidente della Federazione italiana giuoco calcio, il dottor Giancarlo Abete, impegnato com'è in un lavoro ancor più complesso, difficile, articolato. articolato. Arrivo rapidamente alle conclusioni, signor Presidente. Noi riteniamo che questo sia un primo importante momento nel rapporto che lo sport italiano deve avere con le realtà parlamentari. Un altro, come il ministro Melandri sa, lo avremo nelle prossime settimane attraverso il dibattito dedicato ai diritti televisivi del calcio, un altro elemento importante, che servirà per comprendere, per capire come questo sport possa ritrovare anche sul piano agonistico una diversa e nuova vitalità. Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento, convinto com'è che il calcio italiano può e deve uscire dal cono d'ombra nel quale è stato confinato nell'ambito di questi ultimi mesi, dalla spirale di incertezze e di inquietudini che lo ha caratterizzato,

intrecciato alla realtà di una civiltà moderna nella quale il rito di una stupida crudeltà finisce per essere un rito che si trasforma in un'occasione domenicale violenta e al tempo stesso inconcepibile. Noi continueremo a lavorare su questo piano. Siamo convinti che questo provvedimento debba rappresentare la pietra angolare di un sistema nuovo attorno al quale costruire per il futuro dinamiche diverse e al tempo stesso sempre più legate all'attualità del calcio italiano, ma siamo anche convinti che se oggi il Parlamento non fosse riuscito a dare questa risposta nell'opinione pubblica nazionale

Ecco perché, con piena convinzione, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento. Senatore Barbato, io l'avevo chiamato per primo. Lei si iscrive per primo e arriva a metà. Voglio fare un patto con l'Aula: noi diamo la parola al senatore Barbato, pure se l'avevamo saltato,

stiamo per esprimere un voto importante su un testo giunto in seconda lettura in questo ramo del Parlamento a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, modifiche sulle quali si è riscontrata positivamente una sostanziale convergenza tra maggioranza e opposizione. Stessa convergenza, anche se diversa nel merito su talune questioni (quale la norma riformulata in termini di obbligo per le società sportive alla partecipazione e ai costi per l'adeguamento degli impianti) si è registrata sulle modifiche utili e necessarie apportate dalle Commissioni 1a e 2a, condivise anche dal Governo. L'Assemblea del Senato, tuttavia, ha scelto di non procedere all'accoglimento dei suddetti emendamenti confidando nell'impegno dell'Esecutivo a sostegno di un'iniziativa legislativa *ad hoc* da approvare nel più breve tempo possibile. è bene infatti che venga approvato definitivamente il testo licenziato dalla Camera per scongiurare definitivamente il rischio della decadenza di un decreto che difficilmente sarebbe giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica. Certamente l'*iter* di questo provvedimento dimostra quanto, in termini concreti, sia delicata la gestione dei rapporti tra i due rami del Parlamento, ma non è questa la sede più opportuna per affrontare la questione, quanto mai attuale nell'eventuale superamento del sistema del bicameralismo perfetto e paritario che, forse giova ricordarlo, attualmente sopravvive solo in Svizzera e in Romania. Ciò che più conta oggi è, come dicevo, la conversione di un decreto per le misure fondamentali che esso contiene sia dal punto di vista delle sanzioni nei confronti dei terribili episodi di violenza che hanno colpito recentemente il mondo del calcio, sia per il messaggio positivo che vuole lanciare che vuole lanciare attraverso l'introduzione, significativamente ricordata anche nel titolo, di norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

*Allegato A* DISEGNO DI LEGGE Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche